affronto gli aspetti critici di questo provvedimento come se la questione di costituzionalità non esistesse,

dell'impedimento legittimo, ai sensi del 420-*ter*. Di particolare importanza per ciò che dirò di qui a pochi minuti sono le ragioni giustificatrici del legittimo impedimento contenute al comma 1 ed estese al comma

funzioni di governo con espresso rinvio agli atti tipici regolamentati - vengono citate le norme

nonché attività coessenziali alle funzioni. Abbiamo quindi una ripartizione tra funzioni e attività preparatorie, consequenziali e coessenziali. Ai sensi del comma 3, il legittimo impedimento è sottoposto a verifica da parte del giudice; siamo pertanto nell'ambito di una disciplina prevista dal nostro codice di procedura penale. Tuttavia, il comma 4 introduce, come già ho detto stamane, un tipo diverso di legittimo impedimento: legittimo impedimento continuativo, disancorato dall'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale,

giustificato l'impedimento continuativo. Qual è la differenza tra il comma 4 e il comma 1? Cambiano le ragioni del legittimo impedimento:

un impedimento continuativo, nel momento in cui si verifica la sommatoria tra atti tipici delle funzioni, attività preparatoria, attività consequenziale e attività coessenziale - e quindi un complesso di attività - non si spiega il legittimo impedimento continuativo collegato esclusivamente alle funzioni tipiche, cioè ad atti specifici indicati dalle leggi. Se fosse stato il contrario vi sarebbe stata una ragionevolezza. Il comma 1 fa riferimento all'impedimento per l'udienza, e in quel caso si poteva giustificare il legittimo impedimento con il compimento contemporaneo di atti tipici, ma inserito il riferimento esclusivamente alle funzioni indicate al comma 4 come giustificazione dell'impedimento continuativo non ha assolutamente ragionevolezza, in quanto non può assumersi che il compimento di atti tipici codificati nelle leggi citate possa rappresentare un impedimento continuativo, non essendo previsto l'impedimento per le attività preparatorie, consequenziali e coessenziali.

il comma 4? Qualora venga eccepito l'impedimento continuativo, il giudice rinvia il processo all'udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. che il rinvio non può essere superiore a sei mesi, ma che il periodo indicato non può essere superiore a sei mesi.

La giustificazione non regge dinanzi al fatto che, pur sussistendo astrattamente un impedimento continuativo eccedente il termine di sei mesi, il termine consentito è soltanto quello di sei mesi,

il legittimo impedimento per infermità mentale. In quel caso, infatti, è vero che è previsto il rinvio di sei mesi,

mentale dell'imputato, sulla sua capacità di partecipare validamente al dibattimento. In quel caso qui no. Quindi, il periodo massimo di impedimento continuativo è di sei mesi e, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi in materia penale o comunque incidenti sulla materia penale, non è possibile un'interpretazione estensiva. Ciò che è scritto è ciò che vale, ossia sei mesi è il massimo periodo di impedimento continuativo. Allora, se è così, non ha fondamento la giustificazione delle ragioni di tutela della serenità dello svolgimento delle funzioni, in quanto

In effetti non è così: si tratta di una norma transitoria eventuale, in quanto l'articolo assume

dall'entrata in vigore di una legge costituzionale e qualora non vi sia una legge costituzionale, comunque essa non può avere una durata superiore a 18 mesi. viene inserita all'articolo 2 una norma temporanea. Noi stiamo derogando alla Costituzione applicando una norma temporanea della durata di 18 mesi,

nel lodo Alfano era previsto che, in caso di sospensione del processo per legittimo impedimento, comunque il giudice poteva compiere gli atti urgenti di cui agli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Si tratta di una categoria di atti tassativamente previsti dal nostro codice.

che possa dimostrare, attraverso la testimonianza di una persona in fin di vita, la propria innocenza. Il disegno di legge in esame non prevede la possibilità di compiere atti urgenti.

Signora Presidente, in via preliminare intendo esprimere la mia più viva protesta per il modo in cui la maggioranza impone la forza dei numeri anche sui tempi sui tempi del confronto, di cui evidentemente ha paura, così violando gravemente il diritto di ogni senatore ad attendere in modo compiuto al suo mandato. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo disegno di legge di iniziativa di alcuni parlamentari della maggioranza, oltre a lasciare sbigottiti per via della pervicacia con cui in questa legislatura si susseguono le leggi *ad personam*, lascia sconcertati per la natura delle norme in esame a cagione della loro palese contrarietà alla Costituzione. Dopo il fallimento decretato dalla Corte costituzionale a proposito del cosiddetto lodo Alfano sulla sostanziale «immunità del Presidente del Consiglio dei ministri», ecco una nuova invenzione il cosiddetto legittimo impedimento! Quasi a dire: non si vuole concedere al Capo del Governo una sorta di immunità-impunità per tutto il periodo in cui è nell'esercizio delle sue funzioni? Bene, allora, nell'interesse della buona governabilità, si dovrà impedire a qualsiasi magistrato di "scomodare" il Presidente, distogliendolo dalle sue funzioni, che devono essere pertanto considerate come preminenti anche rispetto alle funzioni giurisdizionali. Presidente, colleghi, questa premessa contiene i punti essenziali della inconsistenza delle basi giuridiche su cui si fonda la nuova iniziativa legislativa della maggioranza di Governo.

rapporti con il Vaticano) non pare possano occupare seriamente il Presidente e nemmeno i rapporti del Governo con le istituzioni europee; e, ancora, le decisioni di indirizzo politico generale, le politiche intese a rimuovere le discriminazioni, e simili. Questo in sostanza equivale a dire che il legittimo impedimento verrà autocertificato ininterrottamente per tutto il periodo del mandato. se non ci trovassimo nel più alto consesso legislativo, nel Senato della Repubblica, e se non fossimo quindi senatori, potremmo ironizzare e forse anche apprezzare l'astuzia o il susseguirsi degli espedienti dei parlamentari di maggioranza, i quali, pur di soddisfare gli interessi del loro capo, sono pronti e capaci di pensarle tutte, anche quelle, come nel caso di specie, che poi tanto intelligenti ed acute non appaiono. Registriamo quindi un'evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove è sancito il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sotto differenti aspetti. Innanzitutto, v'è da rilevare una paradossale maggiore tutela per i reati extrafunzionali, per i quali verrebbe riconosciuto questo abnorme legittimo impedimento, al contrario di quelli funzionali, verso i quali l'articolo 96 della Costituzione non riconosce alcun privilegio o prerogativa del genere. Non è pensabile, non è organico al nostro sistema giuridico, né costituzionalmente corretto ipotizzare che una prerogativa concessa per reati di minore disvalore non sia poi riconosciuta nei riguardi di reati di supposto maggiore disvalore, quali sono i reati funzionali. Trattandosi di una vera e propria prerogativa, atteso che si tratta di una deroga permanente connessa alle funzioni, non può esservi dubbio alcuno che per introdurla nel nostro ordinamento si imponga il ricorso alla legge di modifica costituzionale. La Corte, difatti, lo ha ribadito di recente nella sentenza n. 262 del 19 ottobre 2009, dove si legge: «deve ribadirsi che nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o il componente di un organo costituzionale, e si alleghi, quale ragione giustificatrice di essa, l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che un tale *ius* singolare, abbia una precisa copertura costituzionale». In realtà, questo obbligo della procedura costituzionale è ben noto ai presentatori del disegno di legge, che ignoranti non lo sono, al punto che con una procedura a dir poco inusuale, definendo in sostanza il testo di legge proposto (legge ponte o a termine), preannunziano in maniera sfacciata il ricorso ad una successiva successiva legge costituzionale che conterrà una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri. Come dire, per ora regoliamo, o risolviamo il problema specifico del nostro Capo, d'urgenza, con una legge ordinaria, una materia che richiede invece una legge di rango costituzionale, prevedendo espressamente che questa poi verrà emessa successivamente. Impudenza, arroganza, non importa: di certo, siamo di fronte ad una ennesima violazione delle fondamentali regole che il legislatore di uno Stato civile, quale dovrebbe essere il nostro, dovrebbe sempre e comunque rispettare. Qualcuno ha sostenuto in questi giorni che la nuova invenzione o il nuovo espediente proposto dalla maggioranza rappresenterebbe un male minore rispetto al cosiddetto processo breve; intanto registriamo che il processo breve va avanti, atteso che quella previsione di legge, oltre a porre nel nulla alcuni processi sensibili o di interesse per il Governo in carica o per il suo capo, determinerebbe una vera e propria strage di processi di cittadini ignari ed estranei agli interessi superiori del *Premier*. Non credo che, almeno dal punto di vista del sistema giuridico e del complessivo impianto istituzionale e costituzionale, tale valutazione possa essere condivisa come male minore. Ed infatti, con una radicale e deleteria innovazione, di cui non v'è precedente nella storia italiana, si sta per varare una legge che dichiaratamente viola la Costituzione, in attesa che la stessa Costituzione, in merito, venga modificata

innanzi tutto vale la pena rammentare che è regola assoluta, ricavabile dall'intero assetto del codice di procedura penale, che una parte non può mai vincolare il giudice all'accoglimento della sua richiesta. Questo vale, ad esempio, in tema di richiesta di ammissione delle prove, di richiesta dei riti speciali, di richiesta di riunione o di separazione dei processi, ed in tutte le altre occasioni che si possono individuare alla semplice lettura degli articoli del codice di rito. Nemmeno il pubblico ministero lo può fare, *a fortiori* l'imputato. Non è ammesso alcun automatismo tra *petitum* e *decisum*, altrimenti verrebbe violato - e verrà violato - il principio per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (beh, in fondo, questo è diritto costituzionale). Se si costruisce un diritto insindacabile al rinvio del processo, siamo in presenza di una richiesta vincolante, che urta contro il predetto principio. Nella stessa logica, il codice di procedura penale non consente ad una parte - nella specie l'imputato - di sottrarre, a sua discrezione, al processo determinato materiale probatorio al quale la parte stessa ha dato causa, come accade a proposito delle dichiarazioni rese dall'imputato durante la fase delle indagini, in presenza del difensore Anche se l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere, quelle dichiarazioni non vanno perse e sono utilizzabili. Insomma vi è un nucleo di beni sottratti alla disponibilità delle parti e tra questi, *in primis*, l'indipendenza e l'autonomia del giudice di fronte alle richieste delle parti stesse. Il vincolo del giudice, se mai, può essere ravvisato quando una parte eccepisca una nullità o comunque l'inosservanza di un comportamento dovuto. Se esse sussistono, il giudice deve accogliere la richiesta. Ma badate: questa è cosa diversa, poiché il giudice non è soggetto alla richiesta, ma alla legge che imponeva comportamenti processuali diversi, e la parte si limita a far rilevare questa violazione. Mi rendo conto che, a questo punto, qualcuno di voi osserverà che, una volta disposto per legge che l'impedimento sussiste in quelle determinate circostanze, questo è, appunto, un comportamento obbligato per legge, ma io ritengo che non sia così. La tutela dell'imputato impedito fa parte del suo diritto al contraddittorio e, come tale, va confermata. Ma l'articolo 420-*ter* dimostra, più che altrove, che la materia è oggetto di un bilanciamento attento e rigoroso rigoroso tra il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione. Infatti, la situazione che impone il rinvio dell'udienza, da un lato, è definita in termini molto stringenti: il verbo "risulta" toglie spazio ad ogni incertezza e fluidità; l'impedimento non solo deve essere "legittimo" (cioè non costruito artificiosamente dall'imputato: ad esempio, un ricovero ospedaliero che poteva benissimo essere effettuato in un altro momento), ma deve produrre una «assoluta impossibilità a comparire». Questo significa che l'esercizio della giurisdizione è considerato, per il il nostro legislatore costituzionale, un valore di rango molto elevato, tanto che all'imputato può correttamente essere richiesto anche un qualche sacrificio, come il superamento di un disagio fisico non gravissimo o l'accantonamento di altre sue esigenze personali non imprescindibili. Dall'altro lato, in questa materia il giudice è particolarmente libero nella sua valutazione. Infatti, mentre in ogni altro caso di risoluzione di un contrasto, il giudice deve esporre i motivi logico-giuridici della sua decisione, in questa occasione (e, salvo errore, solo in questa occasione) il giudice è addirittura svincolato - sia pure nella situazione particolare

Nel caso del legittimo impedimento regolato dal disegno di legge in esame siamo invece di fronte, addirittura, ad una vera e propria prova legale, e per giunta una prova legale costruita dall'imputato (starei per dire: nell'interesse dell'imputato con la "I" maiuscola). Inoltre, la Corte costituzionale ha già chiaramente espresso l'esigenza di un bilanciamento tra i due valori nella nota sentenza risolutiva del conflitto nella causa Previti. Il giudice non può affermare la prevalenza dell'esercizio della giurisdizione e, a rovescio, il Parlamento non può addurre una illimitata prevalenza dell'esigenza del parlamentare. Allora, è vero, si trattava di un membro del Parlamento, mentre qui si tratta di un Capo del Governo o di un Ministro. Ma questo può significare unicamente che il secondo dei due valori avrà un peso ed una considerazione maggiore, non che annullerà del tutto il primo. E quando si deve operare un bilanciamento, la valutazione non può spettare legge potrà indicare dei parametri da tenere in particolare considerazione, ma non potrà sostituirsi al medesimo. Questo ribadisce in maniera inequivocabile l'illiceità di una prova legale. E voi, colleghi, voi, magistrati, voi, avvocati valenti, non avete alcuna possibilità di contraddire contraddire queste affermazioni, perché sono scritte a caratteri cubitali nel nostro sistema giuridico e nella nostra Costituzione. Voi, però, in maniera pervicace andate avanti perché intendete raggiungere un obiettivo che se, politicamente, vi potrà ripagare, dal punto di vista della storia del Paese, degli equilibri e del rispetto del valore della civiltà giuridica, vi sta facendo ammazzare la Costituzione! Molto opportuno è inoltre considerare che il testo al nostro esame sancisce una presunzione assoluta di impedimento, facendo rinvio ad una serie di norme che descrivono quali sono le attribuzioni del Presidente del Consiglio. E sta bene. Ma queste disposizioni non dicono che tali attribuzioni rappresentano un *continuum* nell'esistenza del Capo del Governo. Dicono semplicemente che, tra i compiti del Capo del Governo,

Questo obbliga a ritenere che non basterà dire che il Capo del Governo è impegnato da una di quelle attività, ma che l'impedimento si manifesta proprio nel giorno dell'udienza, e si esprime «in modo continuativo» (come si legge con tanti interrogativi sulla veridicità dell'attestazione, qualora poi si scopra che il *Premier* quel giorno è andato ad inaugurare una parrocchia o una strada; e con alcuni dubbi sulla possibilità di ravvisare un falso in atto pubblico, posto che sarà la Presidenza del Consiglio a redigere l'attestazione. Badate, dove stiamo andando! Abbiamo constatato che la normativa processuale vigente in materia di impedimento è caratterizzata da un elevato rispetto del valore dell'esercizio della giurisdizione e che la nuova norma non solo entra in tensione molto forte con esso, ma rappresenta una deroga, la quale, secondo le pronunce della Corte, deve essere solidamente giustificata. Entrano allora in campo le due pronunce

comune a tutti gli imputati, ma una prerogativa specifica di alcuni soggetti, titolari di alte cariche pubbliche. È importante notare che il disegno di legge in questione ne dà atto a sua volta in modo esplicito, là dove dichiara formalmente che il fine del disegno è quello di consentire badate - ai vari soggetti il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite. Dunque, non stiamo parlando, cari colleghi, di diritto di difesa, ma di prerogative connesse ad una funzione. Qui, allora, entra in campo l'altra pronuncia, la n. 24 del 2004 sul lodo Schifani. che la sospensione allora introdotta creava «un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione»; che la differenziazione non può essere di per sé esclusa, poiché «situazioni diverse possono implicare differenti normative»; che in tal caso aveva «decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione

funzione pubblica in discorso. Quali sono questi valori? La Corte ne elencò parecchi: il diritto di difesa dell'imputato, privo della facoltà di rinunciare alla sospensione (oggi superato); il diritto della parte civile (oggi ben presente, perché la reiterazione eventuale delle richieste di rinvio non si accompagna neppure a quella moderata compensazione costituita dalla possibilità di trasferire l'azione in sede civile); i tempi del processo, che, sebbene di fronte ad una dilazione che non è indefinita sono tuttavia notevolmente allungati; e soprattutto il «principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione». L'impedire drasticamente al giudice di tenerne conto costituisce una presunzione *iuris et de iure* di prevalenza delle funzioni pubbliche, che urta contro i principi contenuti nella Costituzione. L'esigenza di contemperare è pretesa espressa dalla Corte. Sulla base di queste considerazioni sarebbe auspicabile - nonostante tutto io continuo a sperare ed a sognare - che almeno qualcuno dei colleghi della maggioranza prendesse in considerazione di fare prevalere, almeno in questo momento così delicato per il Paese, la ragione ed il diritto rispetto agli interessi di una sola persona. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è dall'inizio della legislatura che questa Aula è costantemente umiliata dalla necessità di occuparsi di fatti triviali, di processi triviali, per motivi abbietti, che riguardano il Presidente del Consiglio. Siamo inchiodati qui, mentre la società aspetterebbe da noi parole risolutive su problemi fondamentali, ad occuparci solo dei suoi processi e soprattutto del modo di farlo uscire dai processi. Che la legge sia incostituzionale e che contenga numerosi conflitti di interesse e che sia arruffata sotto il profilo stilistico lo ha già dimostrato *ad* *abundantiam* il mio collega Li Gotti, molto meglio di quanto potrei fare io: quindi, non sto nemmeno a ripetere cose di questo tipo. Al giudice è sottratta la materia. Abbiamo una legge distorta e distorcente, ma l'aspetto fondamentale che voglio evidenziare in questa sede nei pochi minuti che mi spettano, e che è impossibile rinunciare a comparare ciò che noi siamo costretti a fare qui con i sinistri scricchiolii che vengono da certe zone della società fuori dall'Aula. Gli organi di stampa, anche insospettabili, hanno raccontato che solo l'altro giorno il Presidente del Consiglio si è permesso di minacciare il Presidente della Repubblica: in nome di che cosa? Io sono eletto dal popolo, tu no, quindi fai come voglio io: questa la logica terribile che esprimono tali leggi. Tutto si deve fare, tutto si deve operare e tutto si deve distorcere nella legge italiana perché lui è l'eletto dal popolo e quindi è sciolto dal vincolo delle leggi e supera ogni confine. Questo è assolutamente inaccettabile e già di per sé rappresenta una perfetta esemplificazione della distorsione cui si sottoporrà la Costituzione - ora c'è già l'anticipo quando si oserà, se mai si oserà, stabilire che il vertice del potere politico deve essere eletto direttamente dal popolo. Cosa ci aspetta? Ci aspetta subito l'atto di sopraffazione di prepotenza di un individuo che, pensando di essere eletto direttamente dal popolo, si prende qualsiasi licenza. *(Commenti dal Gruppo PdL).* Berlusconi non è eletto direttamente dal popolo! Berlusconi è eletto da una legge infame e sbagliata che aveva l'artificio iconografico per cui il nome del Presidente era scritto nel tondo del simbolo.

che rappresenta la perfezione e l'anomalia istituzionale che sarà studiata nei prossimi decenni, perché ciò che accade in questa Aula diventerà materia di studio per l'orrore istituzionale che è maturato dentro le Assemblee elettive.

però siamo convinti che provvedimenti triviali da questa Aula non ne siano mai usciti.

si prendono i voti, si vincono le elezioni, si va al Governo e si cambia la legge.

irrisorio: 239 no a fronte di 316 sì. È stata definita la temporaneità di questo provvedimento;

del Consiglio dei ministri. È stato fatto un gran can-can per far cadere e mettere nel nulla il lodo Alfano che, tutto sommato, era una buona norma era una buona norma che stabiliva che l'attività di governo non avrebbe dovuto essere soggetta a strumentalizzazioni e che per tutta e che per tutta la legislatura si sarebbero accantonati i provvedimenti che toccavano le più alte cariche dello Stato senza nessuno sconto, perché alla fine della legislatura si sarebbero celebrati celebrati i processi e non sarebbe decorso alcun termine di prescrizione e nessun tipo di abbuono. Quando la Consulta

D'altronde, il legittimo impedimento non è una norma avulsa dal nostro sistema; non è un istituto nuovo, ma abbastanza noto: 420-*ter* del codice di procedura penale stabilisce che ogni singolo imputato può invocare il legittimo impedimento e chiedere, pertanto, un rinvio di quella particolare udienza. Addirittura, il giudice può rilevare d'ufficio il legittimo impedimento quando, a suo parere, appaia probabile che l'assenza dell'imputato dipenda dall'assoluta impossibilità a comparire. Che cosa fa in questo caso il giudice? Quello che prevede questa norma: rinvia e comunica all'imputato la data della nuova

sembra che il potere giudiziario non abbia mai preteso ingerenze da parte del potere politico e del potere esecutivo, al punto che fin dall'inizio si è pensato ad una struttura che rendesse veramente indipendenti e autonomi i poteri. Il Consiglio superiore della magistratura è servito sostanzialmente per tenere al riparo gli organi giudicanti da

seguente domanda: è legittimo perseguire la protezione dello svolgimento di funzioni costituzionali e di governo? Tali funzioni sono o no meritevoli di tutela,

Presidente, ancora una volta debbo esprimere il mio disagio nel dovermi pronunciare su un disegno di legge la cui palese incostituzionalità renderebbe inutile qualsiasi osservazione di carattere giuridico.

la Corte costituzionale si pronunzia, dopo di che si grida al complotto. Questa è una prassi a cui stiamo assistendo costantemente e devo dire che lascia sconcertati non solo i parlamentari, ma anche i cittadini italiani. *Repetita non iuvant*, perché il Governo ha una fatale tendenza a reiterare, con una dolosa preordinazione, gli stessi, gravissimi errori: distorcere la legge, in violazione della Costituzione e in danno dei cittadini tutti, per favorire i personalissimi interessi dei soliti noti (in questo caso, al *Premier* abbiamo aggiunto anche i Ministri).

del tutto analoga alla prima, tenendo in non cale le proteste delle opposizioni, basate su ragioni coincidenti con quelle su cui si è fondata l'ennesima declaratoria di illegittimità da parte della sentenza n. 262 del 2009 della Consulta. come nulla fosse, la maggioranza intende approvare un disegno di legge (ancora una volta ordinaria) che, in violazione della Costituzione e del giudicato costituzionale, ripropone - ancorché sotto la diversa veste del "legittimo impedimento" - la stessa forma di immunità che dal 2003 si tenta di introdurre. Con l'aggravante che stavolta non si tratta di "proteggere" le sole quattro più alte cariche dello Stato, ma una categoria molto più estesa di figure istituzionali: l'intero collegio del Consiglio dei ministri. Dell'incostituzionalità di una

In quella pronuncia, nel ritenere inammissibile la tesi della parte privata volta a individuare la finalità della legge nel garantire il diritto di difesa del titolare delle quattro alte cariche, assimilando così la prerogativa prevista a una sorta di presunzione assoluta di legittimo impedimento, si afferma infatti che "il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale e non sarebbe stata necessaria la norma denunciata per tutelare, sotto tale aspetto, la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all'alta carica da lui rivestita. La sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire disposta ai sensi del codice di rito penale contempera il diritto di difesa con le esigenze dell'esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale (sentenze n. 451 del 2005, n. 391 e n. 39 del 2004 e n. 225 del 2001)". Di più: si precisa che "sarebbe intrinsecamente irragionevole e sproporzionata (...) la previsione di una presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo fatto della titolarità della carica. Tale presunzione *iuris et de iure* impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa.". il disegno di legge in esame realizza esattamente ciò che la Corte ha definito essere inammissibile. Infatti, si riconosce a tutti i membri del Consiglio dei ministri il potere di autocertificarsi un impedimento a comparire in udienza, legittimo *ex lege,* anche per periodi di sei mesi;

costituzionale, sentenza n. 140 del 2003), dichiarato dalla Corte costituzionale necessario al rispetto del principio di leale collaborazione tra organi istituzionali, e che richiede non già un'automatica e generalizzata sospensione del processo ma la fissazione del calendario di udienza secondo modalità compatibili con entrambe le suddette esigenze, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare caso per caso l'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto. Il disegno di legge in esame sancisce invece, in favore dei titolari di cariche di Governo, una presunzione di legittimo impedimento assoluta, automatica e non modulabile nel tempo secondo le esigenze di volta in volta addotte, del tutto incongruente dunque rispetto alla finalità di assicurare il diritto di difesa all'imputato, potendo il previsto termine sospensivo essere sproporzionato sia per eccesso che per difetto, a seconda dei casi, non potendo in alcun modo il giudice valutarne la congruità. In tal modo si realizza non solo un'alterazione del rapporto tra poteri dello Stato a detrimento della magistratura e a favore del Governo, ma si finisce per sottomettere addirittura la funzione giurisdizionale (il cui esercizio è finalizzato alla tutela dei diritti di tutti i cittadini e in primo luogo di quelli delle parti processuali) all'insindacabile arbitrio dell'esecutivo. *Dominus* del processo non sarà più dunque il giudice ma l'organo governativo che certificherà, con decisione insindacabile, la sussistenza di un impedimento a comparire, idoneo a dettare il calendario delle udienze e quindi le modalità di esercizio della giurisdizione, in violazione dell'articolo 101, capoverso, della Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (e non anche al Governo) nonché dei principi del corretto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale delle controparti processuali (in base agli articoli 111 e 24 della Costituzione), le quali saranno vittime di una denegata giustizia in nome del "supremo" interesse all'esercizio del mandato. E ciò stupisce vieppiù se si considera che proprio la maggioranza che oggi vota a favore di questo disegno di legge è giunta, con il disegno di legge sul processo breve, al punto di sacrificare l'accertamento della verità processuale in nome della ragionevole durata del processo, preferendone l'estinzione alla prosecuzione per un tempo ritenuto troppo lungo. Un'ulteriore violazione dei diritti delle vittime e dell'effettività della tutela giurisdizionale deriva dall'assenza di norme che consentano, a processo sospeso, di compiere gli atti urgenti e non rinviabili, come sempre viene previsto nei casi di sospensione del processo. manca del tutto un sistema per impedire che un simile istituto si presti ad indebite strumentalizzazioni ed abusi. Una volta che la Presidenza del Consiglio, con un atto fidefacente, abbia attestato che - ad esempio - nei successivi sei mesi mesi non c'è un sol giorno in cui il Presidente possa partecipare alle udienze - neppure il sabato o la domenica, giorni nei quali il giudice deve essere disposto a tenere udienza, come ha insegnato la Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2001, soprattutto quando si tratta di conciliare i giorni della giustizia con le agende dei titolari delle alte cariche istituzionali - cosa accadrebbe se risultasse che qualcuno di quei 180 giorni sia stato dedicato dal membro del Governo ad altro, ad interessi privati? Si dovrebbe avviare un procedimento per falso ideologico a carico di colui che abbia certificato l'impedimento senza soluzione di continuità, talvolta anche in concorso con il soggetto beneficiario, che peraltro - Presidente o Ministro che sia - avrebbe diritto alla sospensione del giudizio, sempre che un altro funzionario sia disposto a certificare l'impedimento ostativo. Si tratta di delicate implicazioni, foriere di preoccupanti momenti di frizione tra politica e magistratura, tanto più inquietanti se si pensa che - almeno stando all'intenzione palesata dai suoi sostenitori questo disegno di legge vorrebbe essere proprio il primo passo verso il superamento di tale frizione. Dunque l'assenza, nella disciplina in esame, di ogni possibilità per il giudice di compiere la verifica dell'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto e il non essersi limitato il legislatore a differenziare «la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario» - come invece richiesto dalla Corte - dimostra come non di legittimo impedimento si tratti, ma di un'immunità, di una prerogativa costituzionale che mai potrebbe introdursi con legge ordinaria. Chiarisce infatti la Corte, nella citata sentenza, che la disciplina di tali istituti, in quanto «diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato», non può essere alterata dal legislatore ordinario «né *in peius* né *in melius*». Un'ulteriore conferma della natura immunitaria dell'istituto introdotto (pur dissimulato sotto le vesti del legittimo impedimento) si rinviene peraltro nello stesso articolo 2, comma 1, del disegno di legge ove, con una sorta di errore freudiano, si precisa che «le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio», al fine di consentirgli «il sereno svolgimento delle funzioni»; non dunque per tutelare il diritto di difesa del Presidente-imputato, bensì la sua serenità, come significativamente si ripromettevano di fare, attraverso la sospensione automatica dei processi, già il cosiddetto lodo Schifani e il cosiddetto lodo Alfano. D'altra parte, se davvero si fosse avuta a cuore la tutela del diritto di difesa del Presidente del Consiglio ogniqualvolta l'impegnativo svolgimento delle sue funzioni ne comprometta la possibilità di partecipare attivamente nel processo, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno neppure di intervenire: il codice di rito prevede già il diritto al rinvio dell'udienza per tutti gli imputati impossibilitati a parteciparvi. Quanto poi alle maggiori difficoltà che comprensibilmente può incontrare il titolare di un'alta carica istituzionale nel prendere parte al processo, la prassi giudiziaria può e deve farsene carico - come insegna la Corte costituzionale - coordinando le esigenze della giustizia con quelle della politica. Cito al riguardo la Corte costituzionale e precisamente la Tale violazione dei principi costituzionali è vieppiù asseverata dall'intrinseca indeterminatezza delle funzioni il cui esercizio costituisce presunzione *ex lege* di legittimo impedimento. Il riferimento a «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo», meramente certificata dall'organo di appartenenza, si presta infatti a determinare uno stallo del processo che può giungere sino a 18 mesi, anche nei casi in cui la partecipazione all'udienza del titolare di carica governativa non avrebbe in alcun modo rappresentato un *vulnus* all'esercizio del mandato. Dunque, l'introduzione di una simile prerogativa potrebbe ritenersi preclusa finanche al legislatore costituzionale, in quanto non solo incide su un principio supremo dell'ordinamento, quale quello di eguaglianza e pari trattamento rispetto alla giurisdizione sottratto persino alla procedura di revisione secondo la Corte costituzionale (al riguardo cito la sentenza n. 1146 del 1988) - ma deroga a tale principio in maniera assolutamente irragionevole, senza differenziare la posizione processuale del membro del Governo solo per lo stretto necessario. *A fortiori*, una simile disciplina non può essere introdotta certamente con legge ordinaria senza violare l'articolo 138 della Costituzione (come già verificatosi per il lodo Schifani e per il lodo Alfano). Ma l'intrinseca irragionevolezza della disciplina proposta dal disegno di legge può apprezzarsi anche in relazione alla più pregnante tutela così apprestata con legge ordinaria ai processi per reati extra o pre-funzionali (che secondo la sentenza n. 262 del 2009 non possono ritenersi presuntivamente meno gravi di quelli funzionali) rispetto a quanto stabilito dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 per i reati funzionali. Si realizza, infatti, la paradossale conseguenza per cui, a parità di impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio potrebbe ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un processo per reato comune ed essere processato, al contempo, per un reato funzionale. Si aggiunga che, a differenza di quanto avviene per l'appunto con l'articolo 96 della Costituzione, il disegno di legge in esame non opera il bilanciamento tra le esigenze di funzionamento degli organi apicali dello Stato e quelle della giustizia, ma si limita a disporre che queste debbano essere sacrificate a quelle, in violazione degli articoli 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione. Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale si riferisce infatti non solo all'inizio, ma anche alla prosecuzione in giudizio dell'azione, oltre che, naturalmente, alla violazione dell'articolo 138. Si consideri, infine, come la prolungata sospensione del processo introduca un grave fattore gravemente distorsivo delle dinamiche processuali e dei princìpi del corretto processo. In particolare, se il legittimo impedimento viene fatto valere a istruttoria probatoria iniziata o conclusa, il giudice sarà costretto a pronunciare sentenza sulla base dei verbali e di qualche sbiaditissimo ricordo, non propriamente all'insegna dei fondanti principi dell'oralità e concentrazione dibattimentale. Si aggiunga che, probabilmente, alla ripresa del processo sarà estremamente difficile o addirittura precluso (ad esempio, per intervenuta pronuncia a carico di un coimputato) coimputato) comporre il medesimo collegio che aveva istruito il dibattimento prima della sospensione. Così il giudizio che abbia subito una lunga interruzione andrebbe spesso rifatto da capo, ripetendo l'assunzione delle medesime prove a distanza di anni, con il rischio incombente della prescrizione. Considerazione, questa, che vale a dimostrare come la prevista sospensione del decorso della prescrizione (articolo 1, comma 5) sia poco più che una norma manifesto. Se non la prescrizione, sarebbe comunque sempre dietro l'angolo di un processo sospeso la sua irragionevole durata, ancora una volta in violazione dei principi del corretto processo. Ancora, nel caso di concorso di persone nel reato, il processo potrebbe procedere separatamente nei confronti di quanti non possono avvalersi della prerogativa *de qua*. Oltre che violare la Costituzione e i diritti delle parti processuali, questo disegno di legge rischia dunque di minare ulteriormente la legittimazione delle istituzioni e il loro fondamento democratico, con un effetto che andrebbe ben al di là della situazione contingente in cui si sviluppa oggi la crisi della politica.

ho seguito con doveroso interesse le argomentazioni di chi sostiene la necessità di questo provvedimento e con altrettanta doverosa attenzione le ragioni di chi vi si oppone, ma non direi cosa sincera - e non sono solito farlo - se dicessi che le ho seguite con particolare passione o emotività. Infatti, essendo questa un'Assemblea politica e legislativa, non un'accademia né un'aula di tribunale, penso sia doveroso dare un contributo e una risposta, pur giuridicamente consapevole, di di intonazione prettamente politica, senza scadere nelle trivialità del confronto politico alle quali ci ha abituato la temperie che stiamo attualmente vivendo. Certo, se io dovessi replicare al linguaggio, paradossalmente, che mi è simpatico, nella sua rudezza, nella sua franchezza e nella sua intransigenza estremistica del collega Pardi, gli direi che se ci dobbiamo fronteggiare a male parole in maniera così aperta lo possiamo pure fare, in Senato come in piazza. Potrei solo rispondergli che, come con qualunque mezzo si vuole abbattere chi ha ricevuto il voto degli elettori e degli italiani per governare, noi abbiamo il dovere, altrettanto bruscamente e in maniera semplificatoria, di non farvi ammazzare Berlusconi per via giudiziaria. Con questo avrei risposto a battuta con battuta, forse anche efficace - mi lusingo di pensare - ma non avrei risolto i problemi.

Se si è posta questa esigenza di intervenire, e se forze politiche anche esterne alla maggioranza di Governo hanno ritenuto, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento, che vi sia la necessità di mettere mano a questo problema, significa che esso è di un'oggettività innegabile. Se poi c'è perfino chi sostiene la tesi del male minore, e cioè vede in questo provvedimento non l'*optimum* ma tuttavia una misura idonea ad affrontare un'emergenza di carattere costituzionale ed istituzionale e certamente una strada preferibile ad altre che vengono considerate addirittura invece devastanti per l'ordinamento e per il sistema, significa che non stiamo determinando una situazione, ma affrontando una situazione nel modo in cui essa si è posta e nelle conseguenze che ne derivano. Voglio dire ancora, non senza un deliberato accento polemico, ai colleghi del maggiore partito di opposizione, che essi sono liberi naturalmente di affidare, delegare o dare in appalto alla categoria dei magistrati la gestione dei problemi dell'emergenza giustizia in Italia e del confronto politico che intorno ad essa si radica; è legittimo. I parlamentari ben possono provenire dai ranghi della magistratura; è un diritto assolutamente incomprimibile, sempre che si mantenga nella correttezza politica di cui pure si discute e si recrimina in questi giorni. Possono farlo, ma tuttavia non possono ignorare la situazione di profondo discredito che una parte della magistratura sta determinando in capo ad uno dei poteri costituzionali della nostra Repubblica, che è appunto il potere giudiziario. E se oggi le rilevazioni danno in flessione il tasso di fiducia nei confronti degli organismi politici o delle istituzioni parlamentari, spero che qualcuno non ignorerà che quella che era una fiducia alta nel presidio della magistratura, che si registrava in tutti i sondaggi negli anni e nei decenni passati, oggi è in caduta libera allo stesso modo, se non in misura addirittura più allarmante.

-ma non è la soluzione dei problemi, anzi incancrenisce ed avvelena i rapporti politici nei quali si calano provvedimenti come questo. Il collega Li Gotti, che sicuramente è stato uno dei più oltranzisti nel criticare questo provvedimento, ciò nondimeno ci ha dato atto che se tutto si limitasse ai primi tre commi dell'articolo 1 alla fine il provvedimento sarebbe quasi accettabile o "transitabile" - non voglio male interpretarlo tuttavia radica le sue critiche soprattutto sul comma 4, oltre che sui successivi, non tenendo presente che in questo caso il vero problema politico, onorevoli senatori, è quello di trovare l'equilibrio tra due esigenze tra due esigenze che i giuristi avvertono e che i legislatori devono avvertire, ma soprattutto i cittadini sentono profondamente. Faccio riferimento ad che i processi, anche a carico del capo del Governo o dei Ministri o di chiunque altro rivesta importanti funzioni pubbliche, pur si facciano e che nessuno sia immune, esente da responsabilità: è un principio sacrosanto, portato avanti dal cittadino prima ancora che da ciascuno di noi.

e di non mettere innanzi scuse o diversivi rispetto a questo incalzante dovere ritenuto tale perfino nei tempi. In una Repubblica, in uno Stato di diritto, che fonda largamente il suo impianto sulla divisione dei poteri, è troppo facile riscontrare invece i debordamenti di questi stessi poteri. E non è ragione di scontata polemica ricordare a ciascuno di noi e a chiunque se ne fosse dimenticato che il potere legislativo e l'investitura di governo traggono il loro fondamento, la scaturigine, da una legittimazione di libere elezioni che a torto vengono svillaneggiate o sottovalutate dal collega Pardi, quando dice che un certo Silvio Berlusconi non è stato eletto dal popolo Tutt'altro: è così, piaccia o non piaccia. Giustamente un egregio collega vi ha ricordato che in democrazia il problema si risolve alla radice vincendo le elezioni, non recriminando sui suoi risultati. Dal punto di vista delle autolimitazioni, il testo contempera queste esigenze, perché proprio la norma stabilisce in sei mesi

distinguere tra le funzioni proprie dettate dalle leggi e le attività preparatorie, consequenziali o coessenziali alle funzioni di governo. Si va piuttosto a spaccare il capello in quattro analizzando il comma 4 cui si parla di funzioni, quasi che la parola stessa non fosse la somma delle incombenze legislativamente stabilite e delle attività preparatorie e consequenziali previste al comma 1. Il limite di sei mesi è dunque un limite che responsabilmente e realisticamente il legislatore si pone, e pone al Governo, ed il Governo accetta che sia imposto alla sua facoltà di attestazione. Non solo, ma il tempo di 18 mesi è un ulteriore autolimite che noi come legislatori, ed il Governo ben accettandolo e dovendolo rispettare, impone alla straordinarietà di questa norma. Concludo dicendo che è tempo - ed è considerazione politica che mi sembra in qualche modo dovrebbe tutti coinvolgerci, in questi giorni, settimane ed ore in cui si pensa di poter giocare con la democrazia su un codicillo o sui cinque minuti dell'orario, o su altre particolarità formali, degne di rispetto

per produrre norme positive e risolvere problemi, di dedicarsi finalmente a quelli che nei comizi dell'opposizione vengono supposti come temi di cui noi non ci occupiamo e che invece il nostro Governo e la nostra maggioranza rivendicano come un proprio diritto e dovere, vale a dire i problemi dei cittadini

della sanità per tutti, della scuola che prepari, selezioni e formi, di riforme anche costituzionali, che senza spinte demagogiche guardino al modo in cui si devono licenziare norme per uno Stato moderno e funzionale.

cosa della quale pagherebbe il prezzo, non certo una maggioranza legittimata da molte prove elettorali, ma tutto intero il sistema delle nostre istituzioni.

importante trovare un accordo, perché la Commissione parlamentare antimafia, così saggiamente diretta dal presidente Pisanu, questa sera dovrà affrontare problemi quanto mai delicati. Io non posso mancare e, come me, gli altri componenti, ma nessuno di noi intende neanche disertare la Commissione giustizia. Ritengo, pertanto, che si debba trovare trovare una composizione, una soluzione che rispetti i diritti dei parlamentari.

per economia di tempo e per non tediare l'Assemblea, il relatore si richiama direttamente. Il relatore non intende neanche spendere parola alcuna per interventi assolutamente connotati per carenza di contenuti e parimenti assoluta grossolanità di linguaggio.

abbiano adeguatamente fornito replica ai profili più strettamente politici sollevati dall'opposizione. L'unica riflessione che il relatore, sia pure in telegrafica sintesi, intende svolgere in sede di replica in quest'Aula trae spunto da alcune considerazioni, diverse e distinte rispetto a quelle che hanno contraddistinto gli interventi degli altri colleghi sia in Commissione che in Aula, fatte con tono estremamente pacato dal senatore Li Gotti.

questa mattina - troverebbero una loro incoerente cesura nel successivo comma 4 dell'articolo 1

situazioni oggettivamente perimetrate nell'articolo 1. Mi pare opportuno, a tale riguardo, ricordare ancora una volta che la Presidenza del Consiglio è organo dello Stato, terzo rispetto alla persona

certifica ed è soggetto terzo - è quindi assolutamente infondato oltre che inesatto parlare di autocertificazione - emette un atto fidefacente. Ma non è questo il senso della replica. Il ragionamento che mi pare opportuno sviluppare, perché porta coerentemente a conclusioni assolutamente diverse e distinte rispetto a quelle del collega Li Gotti, è

è corretto, a maggior ragione nella premessa dell'assoluta terzietà dell'organo che in questo caso svolge una funzione fidefacente nella sua certificazione, occorre vedere cosa si soltanto la razionalizzazione di ciò che il medesimo organo, ovvero la Presidenza del Consiglio, dovrebbe fare per certificare ogni singola situazione che di per sé, nei commi 1, 2 e 3, determinerebbe in modo conferente e coerente un legittimo impedimento nel momento stesso in cui la Presidenza del Consiglio ha

preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alle funzioni del Governo. Diversamente, introdurremmo una semplice suggestione interpretativa. Quindi, nel momento stesso in cui si ha cognizione

la frammentazione e la ripetizione inutile di una serie di certificazioni che dovrebbero susseguirsi l'una all'altra senza soluzione di continuità, le attesta cumulativamente.

ad attestarne semplicemente l'entità e l'importanza ai fini della legittimità dell'impedimento, con un intervento interpretativo del legislatore che riguardando un istituto di carattere ordinario non può essere fatto

Concludendo, il relatore non può che riportarsi alle osservazioni, riflessioni e conclusioni della propria relazione introduttiva. Signor Presidente, credo che alcune osservazioni in relazione alla discussione generale debbano essere effettuate, perché con questo disegno di legge vengono introdotti dei meccanismi di squilibrio istituzionale all'interno del sistema processuale. Questo era uno dei punti fondamentali che avevamo segnalato con i nostri interventi, avevamo segnalato in particolare che, a seguito di giurisprudenza di merito ordinaria, della prassi giudiziaria e soprattutto grazie all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 2001, era stato segnalato il limite del confronto tra potere politico e funzione giurisdizionale ed era stato creato un meccanismo equilibrato, che adesso, con queste norme, rischia di saltare completamente. Quindi, ciò che si definisce uno stato di tensione o di conflitto tra funzioni e poteri rischia di essere oltremodo aggravato. Credo che questa sia una situazione facilmente osservabile, sol che si pensi che tutti i casi della storia recente, ma anche meno recente d'Italia hanno dato modo di verificare come soltanto in questo caso ci sia una pretesa di rottura dell'ordinamento e dell'ordine costituzionale, nel tentativo di creare una situazione di prerogativa a favore del Presidente del Consiglio dei ministri. Il relatore Mugnai, nella sua esposizione, ha motivato ulteriormente e ha richiamato, anche in sede di replica, uno degli aspetti di questa normativa, dicendo che il Governo e la maggioranza ritengono essenziale un intervento del legislatore su questa materia. Come Partito Democratico siamo invece fortemente convinti che in materia di giustizia ci sia ben altro di essenziale: le riforme necessarie sono state già ricordate così come l'accelerazione dei tempi. Questo insieme Questo insieme di norme sembra quasi - utilizzo un'espressione della collega senatrice Incostante - un *prêt-à-porter.* Significa che laddove c'è bisogno di qualcosa, di un modellino, di intervenire, si utilizza uno strumento che possa essere utile al fabbisogno momentaneo e specifico. Ed ora ci viene indicato come altro elemento fondamentale di questo panorama istituzionale un concetto che veramente non abbiamo mai avuto occasione né di leggere né di studiare in alcun testo di diritto. E, quindi, assume una connotazione di principio generale dell'ordinamento la serenità del Presidente del Consiglio dei ministri. A noi sembra questa un'assurdità logica e giuridica e sembrerebbe quasi uno schema protettivo a favore di persone, o di una persona, quasi che fosse - non lo credo - un *minus habens* che abbia bisogno di uno schema di tal genere. Credo che invece istituti quali questo del legittimo impedimento sarebbe possibile rafforzarli, prevedendo però delle norme a tutela di tutte le parti processuali non soltanto di una limitatissima categoria di parti processuali, e nel riconoscimento delle funzioni e dei doveri del giudice. Ma ci sono alcune altre osservazioni che sono state formulate in quest'Aula, dal relatore

dicendo «presunta» violazione dell'articolo 3, «troppo spesso invocata, sì da apparire abusata». Ora, signor Presidente, signori del Governo e della maggioranza, non ci stancheremo mai di ricorrere all'articolo 3 della Costituzione e non abuseremo mai di questo articolo, perché riteniamo che il principio di uguaglianza di tutti cittadini di fronte alla legge e di fronte alla giurisdizione sia un principio costituzionale addirittura sovraordinato e che non debba aversi paura di ricorrere troppo spesso ad un principio di tal genere. Ma c'è un altro punto,

una confessione di recidiva preventiva dice che nulla osta a che si possa procedere a nuovamente interpretare con legge ordinaria l'ambito applicativo dell'articolo Ora, a parte l'elogio del lodo Alfano fatto dal senatore Divina in quest'Aula, noi riteniamo che ricorsi di questo tipo a sistemi di recidiva dimostrino - ovviamente, con rispetto per la persona - quasi una faccia tosta istituzionale, un richiamo alla legge del più forte e un abbandono dei concetti richiamati dalla nostra Carta costituzionale. Non bisogna dimenticare in quest'Aula che il lodo Alfano è stato sonoramente bocciato dalla Corte costituzionale, così come è stato sonoramente bocciato il Ministro della giustizia che su questo tema continua a riproporre le stesse tematiche. Noi riteniamo che non sia possibile ricorrere, su materie così delicate, alla legge del più forte e alla legge dei numeri, perché la democrazia costituzionale è un'altra cosa. Quindi, per questo motivo noi continueremo a riproporre, con i nostri emendamenti, un'impostazione completamente diversa rispetto al gioco della maggioranza e del Governo, che vuole esclusivamente tutelare una sola persona rispetto ai suoi specifici processi.

in materia di impedimento a comparire in udienza, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. La discussione generale unica sul complesso delle due fiducie inizierà immediatamente e si protrarrà fino alla conclusione della seduta di stasera, già fissata per le ore 21.

Per la discussione generale i tempi sono stati nuovamente ripartiti tra i Gruppi secondo lo schema che leggerò, avendo particolare riguardo alle richieste dei Gruppi di opposizione. Le due chiame sulla fiducia avranno luogo domani pomeriggio, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18. Seguiranno, a partire dalle ore 19, le dichiarazioni di voto al fine di consentire il voto finale entro le ore 21 di domani. La Presidenza si riserva di comunicare all'Assemblea l'eventualità della trasmissione diretta televisiva per le dichiarazioni di voto, ove così concordato tra i Gruppi. In attesa del voto di fiducia, le Commissioni potranno convocarsi, fatte salve diverse decisioni assunte all'unanimità dai rispettivi Uffici di Presidenza, per il solo esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di pareri su atti del Governo. In via del tutto eccezionale, la Presidenza ha invitato il Presidente della Commissione giustizia a sospendere l'esame del decreto-legge al suo esame fino al voto di fiducia.

il modo inconsueto con cui viene chiesto il voto di fiducia su un provvedimento che è di squisita ed esclusiva origine parlamentare, dal momento che né un disegno di legge né un maxiemendamento che raccolga

E questo per una ragione molto semplice: quando si pone il voto di fiducia su un provvedimento di esclusiva origine parlamentare, è ovvio che il Governo investa la propria responsabilità su quel provvedimento elevandolo, come ci insegnano la Costituzione e la dottrina, a elemento essenziale del proprio programma di governo. Poiché il il punto del legittimo impedimento non è previsto nel programma di governo con il quale il presidente Berlusconi è diventato Presidente del Consiglio, occorrerà che il presidente Berlusconi venga qui a spiegarci le ragioni per le quali individua nel legittimo impedimento, in un testo - lo ripeto - di esclusiva provenienza parlamentare, un punto essenziale e, anzi direi, in questo contesto, in questa Italia e in questo momento, il punto essenziale di attuazione del proprio programma.

e riguardava una normativa in materia di consiglio d'amministrazione della RAI; un altro risale alla XII legislatura e riguardava il Governo Dini, che pose la questione di fiducia su un provvedimento in materia di servizi di pubblica utilità. Ora, al di là del fatto che ciascuno di noi è pianamente oltre che pienamente in grado di rendersi conto che l'oggetto sul quale si poneva la questione di fiducia era ben altro, ciascuno di voi sa molto meglio di me che si trattava di due Governi tecnici, e sa altrettanto bene che i Governi tecnici hanno come propria caratteristica quella di aggiornare continuamente il programma. Proprio per essere Governi tecnici, infatti, essi non si presentano al voto della Camera con un programma, bensì vengono chiamati a rivestire le funzioni di governo con un programma che si compone di volta in volta, e molto spesso con una collaborazione del Parlamento e delle forze rappresentate in Parlamento assai più cospicua di quanto non accada con un Governo espresso da una maggioranza uscita dalle elezioni. Il ministro Vito si era impegnato a riferirci sulla disponibilità del Presidente del Consiglio all'inizio della seduta di oggi, ma non lo vedo presente. questa ragione, signor Presidente, come peraltro ho preannunciato in Conferenza dei Capigruppo, noi non crediamo che la discussione generale possa iniziare, se prima non avremo notizia dal ministro Vito circa la presenza o meno in quest'Aula del Presidente del Consiglio. Presidente, come ho precisato anche nel corso della Conferenza dei Capigruppo, noi riteniamo la

Quindi, è non buona cosa, ma obbligatorio che il Presidente del Consiglio venga a spiegarci le ragioni dell'urgenza che lo hanno portato a richiedere la fiducia in pieno conflitto di interessi.

e ci dia le sue ragioni, se ne ha. Altrimenti la sua assenza significherà che la sua politica è senza contenuti ed è esercitata solo nell'interesse personale, non certo degli italiani!

discutere serenamente di tale provvedimento e anche di un percorso che fosse, per quanto possibile, in linea con le decisioni della Corte costituzionale in materia. Mi auguro che questo cambio di passo, di strategia e di iniziativa

alle questioni che attengono ai titoli di ammissione dei componenti di questa Camera, e così via. Quello che stiamo cercando di chiedere,

è una vostra libera scelta: non la condividiamo, non la rispettiamo, però credo sia una scelta che debba almeno avere il crisma della trasparenza rispetto a chi vi ha votato. In caso

aderiamo alla richiesta degli altri colleghi di opposizione di avere qui presente il Presidente del Consiglio: credo sia il minimo indispensabile per poter capire che cosa stia succedendo in merito a tale vicenda. Soprattutto, credo sia onesto e leale nei confronti dei cittadini che il Governo spieghi che cosa è cambiato nella sua agenda delle priorità anche rispetto al tema della riforma della giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra francamente che ci si stia nascondendo dietro qualche formalismo eccessivo.

innesca. Questo provvedimento, infatti, è nato nell'altro ramo del Parlamento per iniziativa di un Gruppo dell'opposizione che ora chiede meravigliato e sconcertato cosa sia cambiato. Quali fossero le urgenze al cospetto di quello che è accaduto nel Paese ce lo siamo ricordati fino al 13 dicembre; dopodiché è stata eretta una cortina fumogena e si è fatto finta che che quelle cose non fossero mai accadute, che gli atti di disponibilità e di signorilità e le ricerche di contatto per creare un clima differente nel quale tutti potessero ragionare non fossero esistiti.

Di fronte ad una situazione di questo tipo, ritengo che ogni Governo e ogni Esecutivo, tenendo conto delle sue priorità, abbia la possibilità di contemperare l'etica della convinzione del suo programma con l'etica della responsabilità. Una richiesta, come quella che è stata formulata oggi, nasce anche da questa conciliazione di esigenze. Non mi pare che sia impossibile comprenderlo per chiunque abbia un po' di buona coscienza e sappia quali sono le dinamiche parlamentari. Avevamo 1.780 emendamenti.

«Scipione Ammirato» di Lecce, che salutiamo. Rispondendo a tutti, sapete bene, perché siete tutti parlamentari e conoscete il nostro Regolamento e la nostra Costituzione,

l'opposizione ha chiesto la presenza del Presidente del Consiglio: si tratta di una richiesta che abbiamo girato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ancora non ci ha dato notizia.

L'arroganza è di chi pone il voto di fiducia su un provvedimento di origine parlamentare perché non vuole stare seduto in quest'Aula due giorni a fare il suo dovere, che è quello di votare gli emendamenti dell'opposizione ascoltandone le motivazioni. Non vorrei ricordarle che nella scorsa legislatura un Gruppo che aveva un voto di maggioranza fece 1.740 votazioni sulla finanziaria per dare la possibilità ai colleghi dell'opposizione di spiegare le loro ragioni. Altro che arroganza! Voi ne siete maestri: di arroganza, prepotenza e oltraggio alla Costituzione! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti

continuare a sostenere la nostra richiesta che il Presidente del Consiglio venga in quest'Aula. Ha dichiarato la Giunta per il Regolamento: «Alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbia posto la questione di fiducia si applicano, secondo la prassi costante e non contestata, le norme generali relative alla disciplina della discussione, nonché quelle che regolano l'organizzazione dei lavori». Senatore Quagliariello, francamente non vedo nella nostra richiesta e in questo richiamo al Regolamento alcuna pretesa arrogante, se non la difesa cocciuta e determinata delle prerogative del Senato, non delle opposizioni. Dovrebbe essere suo interesse, senatore Quagliariello, dopo che, per ragioni che non so a che cosa ricondurre,

non ho mai, in nessun momento, pensato di poter mettere la mia firma sotto nessuna norma che anche lontanamente assomigliasse al legittimo impedimento, sono qui scevra da colpe precedenti. E con me se la può pigliare con tutto il gusto che le

Ciò che non va è l'arroganza di pensare di prendere in giro anche i Gruppi di opposizione: questo è quello di cui voi dovreste ogni tanto - non dico sempre, anche poco poco - vergognarvi.

Colleghi, vorrei ribadire un concetto, una mia considerazione. La richiesta della presidente Finocchiaro in merito alla presenza del Presidente del Consiglio è una richiesta politicamente legittima: non ci trovo niente di strano. nessun rimedio parlamentare è previsto per la obbligatorietà della presenza del Presidente del Consiglio. Il richiamo fatto dalla presidente Finocchiaro alla ordinarietà della legislazione per la presenza del Governo - lei mi insegna è disciplinato organicamente dalla facoltà del Governo di farsi rappresentare in Aula. Tante volte, dai banchi sia della maggioranza che dell'opposizione, ho visto chi mi ha preceduto su questo autorevole scanno replicare che il Governo era rappresentato. Governo era rappresentato. Consentitemi soltanto una mia personale considerazione, che può essere smentita anche dall'impedimento del Ministro della giustizia: condivido l'opportunità ventilata dal presidente D'Alia della presenza del Ministro della giustizia, ma sono valutazioni che devono confrontarsi poi con l'obiettiva disponibilità dei rappresentanti del Governo. Fermo restando che quella della presidente Finocchiaro è una proposta di carattere politico, legittima perché ognuno esplica il suo ruolo e quindi la presidente Finocchiaro manifesta la sua idea, a me sta naturalmente applicare le regole e le regole, le conosciamo tutti, non impongono proceduralmente, né a me né a nessuno, di pretendere la presenza del Presidente del Consiglio. La possiamo auspicare, l'opposizione l'ha chiesta, aspettiamo che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ci faccia avere una risposta.

però questo argomento lo ritengo chiuso. un ordine necessario, siamo a chiederle di chiudere la seduta odierna e di riconvocarci domani mattina, quando lei avrà avuto modo di sapere dal Governo sapere dal Governo quale Ministro è libero di poter partecipare e dare così decoro a questa discussione.

non capisco per quale motivo devo sospendere. Non vi sono iscritti a parlare del suo Gruppo,

vorrei sottoporle un ulteriore profilo regolamentare, fermo restando quanto è stato detto così efficacemente dalla presidente Finocchiaro e dagli altri Presidenti dei Gruppi: Gruppi: la questione di fiducia, signor Presidente, secondo il nostro Regolamento, deve essere motivata.

abbiamo la necessità inderogabile, per rispetto del Regolamento, di conoscere la ragione per la quale il Governo ha inteso porre la questione di fiducia, anche eventualmente - è questa la richiesta ulteriore - acquisendo il verbale del Consiglio dei ministri. Si tratta di un atto che può e deve essere reso disponibile al Senato

risultava essere stata autorizzata dal Consiglio dei ministri: presentammo una normale interrogazione e, dopo molti mesi, ci fu risposto che, nonostante quanto alcuni Ministri avevano